con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Senatori, è con sentimenti di affettuosa commozione

Valerio Ferrara è stato un instancabile protagonista della vita sociale, economica e istituzionale di quei territori, oltre che un sensibile interprete e un instancabile difensore delle loro peculiarità. Persona di vivace intelligenza, imprenditore, sindaco, amministratore locale e componente di questa Assemblea per ben tre legislature, Valerio Carrara ha sempre vissuto ogni sua esperienza nelle istituzioni e nella società con grande passione, libertà di pensiero, concretezza e pragmatismo. Il suo era un carattere aperto e dialogante, lo ricordo bene, ma non per questo meno battagliero. Forte era il suo rispetto per le istituzioni, specie quelle parlamentari, come ebbe modo di dimostrare anche presiedendo, con alto senso di responsabilità, imparzialità, competenza e rigore, la Commissione difesa del Senato durante la XIV legislatura, conquistandosi la stima e l'apprezzamento di tutti i Gruppi parlamentari. Grande era l'attenzione che metteva in ogni dettaglio dell'attività parlamentare: dalla scrittura degli emendamenti alla cura degli interventi, sempre puntuali ed efficaci. Valerio Carrara perdiamo un amico, un collega di tante battaglie parlamentari, un politico dal forte tratto umano, garbato, ironico e con una fede incrollabile nelle proprie idee, ma sempre pronto al confronto e alla dialettica costruttiva, senza preconcetti o pregiudizi, nell'interesse dei cittadini e dei territori. Nel rinnovare pertanto alla moglie Ornella, ai figli, ai nipoti e ai familiari del senatore Valerio Carrara il mio commosso abbraccio e la vicinanza mia e di tutto il Senato, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

*(FIBP-UDC)*. Ringrazio la presidente Casellati per la vicinanza che ha espresso a suo nome e a nome di tutto il Senato e di tutti i senatori, anche nel momento del suffragio e del saluto che abbiamo tributato al senatore Carrara Il senatore Valerio Carrara era un uomo delle istituzioni e un uomo del popolo, un uomo della gente e per la gente, un uomo dedito all'ascolto e al lavoro, un senatore e un sindaco, legislatore e amministratore, Vale per gli amici (lo chiamavamo tutti così). Laureato in farmacia, titolare di diverse attività, senatore per tre legislature, dal 2001 al 2013, dal 2004 in Forza Italia e nel Popolo della Libertà. È stato anche, come è stato ricordato, Presidente della Commissione difesa del Senato, un grande motivo di orgoglio, una carica che assunse con grande senso di responsabilità e di serietà. Stimatissimo sindaco per due mandati del suo paese natale e di vita, quella Oltre Il Colle che abbiamo citato, un territorio di montagna. Amava le sue montagne Valerio, amava le nostre valli bergamasche e per il suo territorio si batteva con impegno e determinazione. Amava la vita, era un uomo appassionato e appassionante, pieno di entusiasmo, di ottimismo, estremamente ironico, dalla brillante intelligenza, sempre pronto all'ascolto, sempre pronto alla condivisione e al consiglio. Pratico e concreto come tutta la gente di montagna, con un cuore grande e una propensione naturale alla socialità più diretta. Quando la scorsa settimana mi hanno chiamata per darmi la brutta notizia della sua scomparsa, sono rimasta davvero senza parole, profondamente dispiaciuta, anche perché era giovane, il senatore Carrara. Il dispiacere è stato grande proprio perché Valerio era l'emblema della vitalità e dell'amore per la vita. appassionato ed appassionante, innamorato della sua montagna, del suo bellissimo paese, si è sempre distinto per l'amore per la sua terra. Appassionato dei suoi cavalli, mi parlava sempre del senso di libertà e di comunione con la natura che provava in sella sia ai suoi cavalli, sia alla sua moto. Appassionato cacciatore di montagna, dove si diventa guardiani dei boschi, e innamorato della sua famiglia, della sua Ornella, dei suoi figli Giorgio e Alessandro, delle sue nuore e dei suoi nipoti. Saluto quindi da bergamasca la sua Oltre Il Colle a cavallo tra Val Brembana, Val Serina e Val Seriana e saluto un uomo appassionato di politica, quella bella, quella dell'impegno, quella del servizio, per rappresentare le istanze di quei piccoli Comuni che sono il cuore del Paese, troppo spesso dimenticati. Al di là della perdita, per le istituzioni e per la politica, di un uomo così brillante e generoso, c'è il dispiacere di aver perso un caro amico, di cui conservo tanti ricordi. Ti saluto, Valerio, in quest'Aula, a nome di tutti i colleghi che ti hanno conosciuto e a nome di tutto il territorio bergamasco. Signor Presidente, dopo il ricordo del senatore Carrara, così ben espresso da lei, Presidente, e dalla senatrice Gallone, desidero aggiungere alcune parole. Valerio è stato senatore per tre legislature ed è stato per dodici anni in questa Aula. Ci arrivò in modo inaspettato, ma seppe interpretare molto bene il suo ruolo di rappresentante dei cittadini in generale e del suo territorio, al quale era così legato, come è stato detto poc'anzi. Ha sempre preso con distacco, ironia e anche autoironia i successi. Il fatto di essere arrivato al ruolo di senatore, per una per una persona che ha sempre avuto la passione della politica e dell'amministrazione del suo territorio, era certamente una grande soddisfazione, così stato eletto per altre due legislature ed essere diventato presidente della Commissione difesa, che condusse con capacità ed equilibrio. Erano certamente grandi successi, ma non cambiarono il suo atteggiamento sorridente e cosciente della della transitorietà di tutti i ruoli ricoperti. Allo stesso modo seppe affrontare con altrettanto distacco le feroci critiche che pure gli vennero mosse in uno dei tanti

sua passione per la natura, per le sue montagne, per il suo Comune, quando è stato eletto sindaco con una grande maggioranza di voti. Ricordo bene che mi disse più volte, essendo passati attraverso vicende mediche e chirurgiche in tempi simili: «Dopo quello che ho passato (io sono stato salvato dai chirurghi in modo quasi miracoloso), tutto quello che viene dopo per me è un grande regalo e sto cercando di goderne, di farne il meglio nella mia vita». nella mia vita». Di qui il suo amore per la famiglia, per le sue montagne e per la natura, nella quale cercava di immergersi più possibile; del resto, abitando in un un paese di montagna, era più facile. L'ho sempre sentito con una grande serenità e cosciente del fatto che doveva davvero assaporare questi anni della sua vita, per quanto lunghi fossero stati. Purtroppo sono terminati alcuni giorni fa, ma sappiamo di aver avuto fra di noi, come amico e come collega, una persona vera, una persona che ha saputo esprimere il sentimento di tanti nostri concittadini che qui abbiamo l'onore di rappresentare. A nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, porgo le condoglianze alla sua famiglia, alla quale era tanto legato, ricordandolo con affetto e portando nei nostri cuori il suo bel ricordo.

Purtroppo, dopo qualche giorno di ricovero in ospedale per problemi di salute, è stato colto improvvisamente da un infarto che l'ha strappato ai suoi affetti più cari e purtroppo non ce l'ha fatta. Valerio era un punto di riferimento per tanti; ha amato profondamente la sua terra e la sua comunità, dimostrando come la politica possa nascere e svilupparsi proprio dai piccoli borghi, senza mai dimenticarsi delle esigenze delle comunità da cui si proviene, anche se l'impegno politico poi si sviluppa su un piano nazionale. Desidero ricordarlo per l'impegno, l'entusiasmo e la fervente passione per la caccia e per la montagna, che lo hanno reso protagonista di tante battaglie a favore del mondo venatorio. Un autentico e autorevole rappresentante della comunità bergamasca, ma anche un autentico e autorevole rappresentante delle istituzioni nazionali. Si è speso sempre per numerosi progetti di sviluppo delle zone montane. A nome del Gruppo Italia Viva-PSI, mi stringo alla famiglia, ai suoi cari e alla sua comunità

Signor Presidente, la ringrazio per le parole che ha utilizzato per ricordare il senatore Carrara. Il mio ricordo del senatore Carrara è quello di un uomo intelligente, ironico, innamorato della sua famiglia, con una grandissima passione per la caccia, per i suoi cavalli, e profondamente legato alla sua, alle nostre montagne e alla terra bergamasca. Valerio Carrara era nato nel 1951, laureato in farmacia lavorava come imprenditore, titolare di diverse attività commerciali ad Oltre Il Colle, il suo paese, la sua comunità. Il suo impegno nelle istituzioni iniziò in età matura, sulla spinta del figlio che lo convinse a candidarsi alle elezioni politiche del 2001, nel collegio senatoriale di Albino. Carrara venne eletto e scelse di iscriversi al Gruppo Misto come esponente unico del Movimento Territorio Lombardo. Nel 2004, come ha ricordato la senatrice Gallone, aderì al Gruppo Forza Italia e in Forza Italia prima e nel PDL poi si svolse il suo impegno nelle successive legislature fino alla Presidenza della Commissione difesa del Senato. Oltre all'impegno parlamentare, dell'esperienza di Valerio Carrara merita essere ricordato l'impegno amministrativo al servizio del suo paese natale e della sua comunità. La scomparsa

La scomparsa prematura del senatore Carrara ha rappresentato una perdita significativa per il mondo politico-istituzionale, in particolare per la politica e le istituzioni bergamasche. Il pensiero pensiero del Gruppo Partito Democratico va alla famiglia del senatore Carrara e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e che con lui hanno collaborato in questi lunghi anni.

Signor Presidente, Valerio Carrara era un uomo legato alla sua terra, alla Val Brembana, al suo paese, Oltre Il Colle, dove ha fatto il sindaco per dieci anni. tredici anni di attività parlamentare non si è mai risparmiato nel fare il bene della gente con passione e nel portare avanti le istanze della montagna e la sua grande passione, la caccia. La caccia lo aveva fatto diventare uno dei più autorevoli riferimenti del mondo venatorio in Parlamento; non a caso, era anche consigliere provinciale della Federazione italiana caccia. In contemporanea ai suoi anni in Senato, ha vissuto il ruolo di sindaco di Oltre Il Colle, dove è stato eletto per due mandati, fino al 2017, carica che lo ha fatto restare vicino alla gente e agli amministratori locali, senza dimenticare le sue origini, quelle della montagna. Era un amante della natura, degli spazi aperti, dei cavalli, dello sport e in particolare dell'enduro, una tradizione molto forte nelle valli bergamasche. Per il suo territorio, per lo sviluppo della Val Brembana, per anni cercò invano di sollecitare la riapertura del casinò di San Pellegrino, proprio per rilanciare il turismo nella valle. Ci lascia un uomo un uomo della montagna, un uomo della sua valle, un uomo che non ha mai perso le sue radici e che vedeva nella politica l'opportunità di dare voce al territorio. Tutto il Gruppo Lega e soprattutto i senatori bergamaschi si uniscono al momento di dolore della famiglia. La ringrazio, quindi, signor Presidente, per le belle parole e mi unisco anche alle parole di tutti i colleghi che mi hanno preceduto.

in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale

parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Stefano Candiani costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sulla vicenda del senatore Giarrusso soltanto per evidenziare l'anomalia che si sta verificando in quest'Aula. Noi stiamo qui, oggi, discutendo se

quello che pensa, non può fare una relazione per difendere se stesso. Tutto questo perché non ha il *super green pass*. Si pensi che gli imputati possono entrare senza avere il *super green pass*; invece, in quest'Aula, che dovrebbe essere il tempio della dialettica e delle contrapposte opinioni, quando si discute se mandare a processo o meno il senatore Giarrusso, al senatore Giarrusso non è consentito entrare. Chi non vede che questa è una torsione intollerabile, che dovrebbe farci vergognare tutti, è in malafede.

ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nei casi in cui la dichiarazione esterna cioè *extramoenia* - del parlamentare alla stampa o sui *social* abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è la sostanziale corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione espressa all'esterno delle Aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale. Queste considerazioni sono correttamente ricordate nella relazione, ma poi paiono dimenticate nelle conclusioni. *(Brusio).* Signor Presidente, non riesco a sentire nemmeno me stesso, quindi se lei potesse cercare di...

Infatti, nel caso di specie, l'atto *extra moenia* è un *post* su Facebook del 24 agosto 2020 e quello *intra moenia* è un'interrogazione del successivo 10 settembre. Ancorché si ravvisi una sostanziale corrispondenza di contenuto, appare chiaro come la dichiarazione interna, ossia l'interrogazione, sia motivata dall'intento di avvalersi dell'insindacabilità e non già l'intervento sui *social* motivato, poi, dall'intento divulgativo di un atto parlamentare compiuto. Con tale motivazione dichiaro il voto contrario di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla proposta conclusiva formulata dal relatore. Spero che almeno le conclusioni siano state percepite. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Io l'ho seguita con attenzione, Presidente, e credo che chi voleva l'abbia potuto fare.

Giarrusso viene chiamato a rispondere per le dichiarazioni pubblicate su una pagina Facebook.

Che il senatore Giarrusso non possa partecipare, come sempre accade, a una discussione che lo riguarda personalmente per questioni del tutto estranee alla alla vita parlamentare è un fatto davvero problematico e dovrebbero farsi delle domande coloro che votano certi provvedimenti che poi si riflettono quasi inevitabilmente sulla dinamica del Senato. seconda considerazione. Noi votiamo a favore dell'insindacabilità perché è una prerogativa del Parlamento a difesa non della persona e neanche del singolo senatore, ma delle Istituzioni. Proprio per questo, però, chi ricopre cariche parlamentari dovrebbe evitare affermazioni, come quella di cui stiamo trattando, che hanno senza dubbio offeso ingiustamente delle persone e i loro familiari. il senso di responsabilità deve essere ricordato. Bisogna ricordare che si hanno giustamente delle prerogative in quanto parlamentari, ma questo deve portare a una grande prudenza prima di fare attacchi personali rispetto ai quali noi, per tutelare le Istituzioni, conseguenze giudiziarie che possono essere molto onerose. Tuttavia - lo ripeto - va richiamato il senso di responsabilità quando si fanno certe affermazioni.

nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

del tribunale di Roma, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, non vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

voglio citare il contenuto di un'intervista del senatore Giarrusso al giornale «La verità» dell'8 giugno 2020. Il sottotitolo dell'intervista recita «Basentini, ex capo del DAP, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?». L'intervista ingenera l'idea che la scarcerazione di Zagaria e di altri 40 rappresentanti di alto livello della criminalità organizzata sarebbe stata determinata dal comportamento del capo del DAP, dottor Basentini, che avrebbe garantito questa scarcerazione emanando appositi provvedimenti amministrativi. Sappiamo bene che tutto è avvenuto nel momento iniziale della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 e che quindi i fatti sono andati certamente in maniera diversa. Si sottolinea inoltre che il senatore Giarrusso non ha fatto presente un dato di fatto e cioè che l'incontro con Zagaria del capo del DAP sarebbe durato soltanto pochi minuti, sarebbe avvenuto alla presenza di diverse persone, tutte identificate, secondo la prassi tenuta in occasione delle visite in carcere del capo del

in cui si parla delle rivolte in carcere e del problema della responsabilità eventuale della gestione degli istituti penitenziari, che non hanno nulla a che vedere con l'accusa nei confronti del capo del DAP che, dopo un colloquio con un 'ndranghetista di rango, avrebbe poi emanato dei provvedimenti a favore di camorristi e di tutti coloro che erano nelle stesse condizioni. Sotto questo profilo non vedo alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare. Per tale motivo

Presidente, anche in questo caso sembra ravvisabile un nesso funzionale tra atti *intra moenia* ed *extra moenia* estremamente flebile. Non sembra infatti essere sufficiente il richiamo all'attività parlamentare contro i cosiddetti impresentabili in linea generale per poter giustificare le affermazioni tramite *social network*, che potrebbero configurare un reato di diffamazione a mezzo stampa. Lo stesso soggetto querelante non risulta essere citato negli atti parlamentari del senatore Giarrusso. Infine, anche il nesso temporale fra i *post* pubblicati e gli atti parlamentari non sembra sussistere, considerando che le interrogazioni cui si fa riferimento sono datate dal 2014

presso il tribunale di Catania, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di

della relazione che lei ha citato. Non evito di sottolineare che, dei tre casi affrontati oggi, questo è probabilmente il più lineare, quindi insistiamo perché la relazione venga approvata.

almeno per chi vuole prestare attenzione - seguisse quali sono i fatti all'origine del procedimento che riguarda il senatore Giarrusso. Egli aveva pubblicato su Facebook offensivi della reputazione della signora Debora Borgese, contenenti le seguenti parole: «Pensate che una nota lingua velenosa catanese, malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia la discendente di Madame de Pompadour», «Una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d'Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie», «Attento alla sfiga»

bile». Io non so cosa c'entri questo con l'attività parlamentare. Non vedo quale nesso ci possa essere tra l'attività di denunzia delle infiltrazioni negli enti locali con dei gratuiti insulti e offese a un cittadino che giustamente ha presentato una querela per diffamazione.

di metafore con personaggi della storia francese, dell'accusa di portare sfortuna. Pur ritenendo il tema delle infiltrazioni mafiose negli enti locali di enorme importanza, credo che tutti noi dovremmo concordare sul principio che le battaglie politiche e la difesa della legalità debbano restare su un piano di scontro anche particolarmente duro, ma non scadere in questo modo. Non vorrei in nessun caso che si scambi la tutela costituzionale del parlamentare con una patente a poter dire qualunque cosa e a offendere chiunque. Con tali motivazioni dichiaro il voto contrario di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla proposta conclusiva formulata dal relatore.

di ritenere che il fatto, per il quale il senatore Mario Michele Giarrusso ha ricevuto un atto di citazione pendente presso il tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione).*

Grazie,

svolgendo un'ispezione parlamentare in un quartiere della città di Catania, ha reso conto di questa sua visita in un video di Facebook in cui denunciava il degrado del quartiere e tutta una serie di problematiche del territorio, all'epoca nella sua veste - credo - di commissario regionale della Lega in Sicilia. Un'associazione ha ritenuto che le sue affermazioni fossero da giudicare diffamatorie lesive di una serie di norme. La Giunta, espletata la procedura prescritta dal Regolamento, sentito il senatore Candiani, ha riscontrato che esistevano delle interrogazioni

queste materie per essersene occupato da Presidente della Giunta - la Giunta ha ritenuto che quel video fosse sostanzialmente coincidente con le attività parlamentari delle interrogazioni il senatore Candiani aveva svolto e quindi ha ritenuto che avesse legittimamente espresso delle opinioni non perseguibili. È per questo che la Giunta ha ritenuto di riconoscere le esimenti. La relazione

nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue

che ha generato una serie di commenti che hanno portato a contestargli il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale,

assimilando le condotte di Candiani a delle condotte tenute dall'onorevole Borghezio, ritenendo che Candiani abbia manifestato le proprie idee fuori dalla sede parlamentare e fuori dai limiti dell'insindacabilità. Tuttavia, devo dire che nel caso di specie, oltre alle interrogazioni parlamentari del senatore Candiani sul tema dell'immigrazione, e di tutte le dichiarazioni *extra moenia* sono in questo caso coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, esistendo una sostanziale coincidenza contenutistica, contenutistica, il senatore Candiani si è limitato a un video che ha dato atto di una situazione drammatica del quartiere San Berillo di Catania, in cui c'era questo fenomeno di immigrazione e non ha espresso opinioni, ma ha solamente commentato la situazione. Ritengo quindi che, al di là delle legittime opinioni politiche differenti sul fenomeno dell'immigrazione, dopo aver visto il filmato all'origine del procedimento penale,

Come abbiamo appena sentito, il senatore Candiani ha girato un video nel quartiere San Berillo a Catania che ha pubblicato a luglio del 2018 sul profilo Facebook e mentre girava il video commentava che il quartiere fosse in stato di degrado, in mano ad immigrati clandestini dediti a tutti i tipi di criminalità. Queste sono affermazioni fatte senza conoscere l'effettiva asserita illegalità e clandestinità di tutte le persone presenti, che invece si muovevano in una situazione del tutto legittima. Nel video non si non si riesce a vedere tutto ciò che Candiani afferma facendo riferimento a clandestinità e criminalità. Inoltre, queste affermazioni hanno generato su Facebook, come si poteva prevedere, una serie di manifestazioni di odio razziale e discriminazione. Ora, il relatore propone di concedere la prerogativa dell'insindacabilità perché ravvisa il requisito del nesso funzionale tra la dichiarazione resa nel video ed una interrogazione firmata anche dal senatore Candiani. L'interrogazione parlamentare cui si riferisce il relatore tocca il tema dell'immigrazione, però in modo generico, riferendosi al piano nazionale ed extranazionale. Pertanto il nesso funzionale tra l'atto *intra moenia*, decisamente generico, e quello *extra moenia*, invece decisamente localistico (perché indica azioni specifiche e determinate) risulta essere estremamente flebile. Inoltre devo evidenziare - come dicevo - che non c'è coerenza fra le dichiarazioni espresse nel video dal senatore Candiani e quanto le immagini mostrano, giacché il contesto dei soggetti videoripresi è assolutamente ordinario Quindi, non c'è nemmeno quel pur flebile nesso funzionale ipotizzato dal relatore per l'applicazione delle prerogative. Sintetizzo molto: questa cosa non la dico solo io, ma la evidenzia e la chiarisce spesso anche la Corte costituzionale, per esempio nella sentenza n. 144 del 2015, secondo la quale non è sufficiente un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale o un mero contesto politico per concedere l'insindacabilità dal giudizio della magistratura. A questo quadro, che è di per sé già chiaro, si aggiunge la visione del MoVimento, che rifiuta l'immunità concessa a ogni costo, solo perché parlamentari, giacché in questo caso appunto il nesso con l'attività non sussiste. Vado alle conclusioni. Brevemente: si vuole concedere l'insindacabilità? Bene, facciamolo, ma facciamolo solo in casi alti, eccezionali, importanti, non in questo, così da rispettare il progetto originario dei nostri Padri costituenti. Non sviliamo la Costituzione; questo antico istituto costituzionale oggi, per come è stato trattato, è ridotto a un privilegio odioso, tipico di chi crede di essere superiore ai normali cittadini. Concludendo, colleghi, il MoVimento 5 Stelle non concede l'immunità e ritiene che questo caso vada chiarito e risolto davanti alla magistratura. Annuncio così il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

esprimere sinteticamente il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore, aggiungendo un aspetto. Nel provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari

usato il fatto che, nei commenti a quanto ha postato su Facebook il senatore Candiani, ci siano state espressioni di odio e così via. Ebbene, direi che bisogna tenere ben distinto ciò che il parlamentare dice (parlamentare o non parlamentare) dalle reazioni che questo può suscitare da parte di chi segue questo *social media*, perché sappiamo bene che nei *social media* basta a volte anche semplicemente dire qualcosa («buongiorno a tutti»)

nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore

senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma,

- la disciplina costituzionale dell'articolo 68 a condotte che nulla hanno a che fare con la legittima libertà di opinione collegata al mandato parlamentare. Non vedo infatti come la rivelazione del segreto d'ufficio, contestata dal tribunale di Modena al senatore Giovanardi, possa configurarsi come un'opinione espressa. espressa. Lo stesso discorso vale per gli altri reati contestati, come la violenza e minaccia a un corpo politico amministrativo o giudiziario. Come si può ritenere che ci sia un nesso funzionale tra i fatti contestati con tali reati e le opinioni comunque espresse dal parlamentare? Per questa ragione, dichiaro il voto contrario di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla relazione del senatore Pillon.

pubblici ufficiali e gli sono contestati diversi reati come la rivelazione del segreto d'ufficio, l'oltraggio e la minaccia, il tutto per tutelare l'impresa Bianchini, esclusa dalla *white list* (un'impresa finita anche sotto processo, tanto che alcuni suoi componenti sono già stati condannati). La relazione del senatore Pillon è volta al riconoscimento della prerogativa per tutti questi pesanti capi di imputazione. fare alcune riflessioni, la prima delle quali è che stiamo parlando di comportamenti posti in atto dall'indagato e non di opinioni espresse. pur non volendo entrare nel merito della rilevanza penale di simili odiose azioni attribuite all'ex senatore Giovanardi, osservo che il relatore tende a confondere la tutela prevista dall'articolo 68 sulle opinioni espresse da un parlamentare con le azioni poste in atto da un parlamentare.

Quindi, questo approccio è foriero di una estensione arbitraria e ingiustificata dell'ambito della insindacabilità delle opinioni a qualsiasi condotta posta in essere dai parlamentari. La prerogativa dell'insindacabilità è volta a tutelare il parlamentare ragionevolmente rispetto a pressioni che sul medesimo possono esercitare altri poteri dello Stato o gruppi di potere esterni. Ebbene, se convenite con me su questo principio, dovete ammettere che nel caso in esame invece è il senatore Giovanardi a fare indebite pressioni sulle attività amministrative e giudiziarie del proprio territorio. Quindi è l'esatto contrario. La Corte costituzionale, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione, nel senso di censurare la delibera parlamentare di insindacabilità, ha rimarcato che la prerogativa parlamentare non può essere estesa fino a comprendere insulti e comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. Allora, è più che lecito estendere questa affermazione della Corte costituzionale a maggior ragione alle minacce. Nel caso in esame, a conforto della mia riflessione, le minacce non possono in alcun modo rappresentare un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, giacché esulano dalla funzione parlamentare, in quanto rivolte direttamente ad organi competenti, per spingerli a modificare i provvedimenti amministrativi sgraditi al parlamentare. Concludo, signor Presidente, dicendo che a questo quadro, già di per sé più che chiaro, si aggiunge il principio che il MoVimento 5 Stelle rifiuta lo stravolgimento dell'articolo 68 della Costituzione. Confermo il mio parere assolutamente contrario alla proposta formulata dal relatore Pillon. In conclusione, ritengo non si debba concedere l'immunità all'ex senatore Giovanardi. Per tutti i motivi esposti, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

che correttamente esaminava la questione e proponeva, su tre capi di imputazione, di stare esattamente a quello che la Costituzione ci attribuisce, ovvero di esprimerci sulle opinioni e dichiarazioni espresse. espresse. È contestato il reato di oltraggio e noi abbiamo fatto una valutazione, votando favorevolmente alla concessione della prerogativa per il reato di oltraggio, riconoscendo il fatto che, comunque, le battaglie del senatore Giovanardi sono note; c'erano comunque dichiarazioni cospicue in Aula. Abbiamo riconosciuto il principio, anche se i toni possono essere esondanti ed eccessivi, difendendo proprio lo spirito e l'intenzione del Costituente di garantire al parlamentare l'attività di denuncia politica e le sue battaglie. Ovviamente non tocca entrare nella condivisione o no delle battaglie. Questo vale anche per il caso precedente del collega Candiani. È ovvio che noi non ci esprimiamo valutando se condividiamo. Il punto è la prerogativa, che garantisce la libertà di denuncia politica. Invece, purtroppo, gli altri due capi di imputazione contestano, vorrei ricordarlo, condotte materiali

decidere noi di cambiare il capo di imputazione, senza che sia stato fatto un processo? Questo è il punto. Io credo che noi, non solo non possiamo, ma non dobbiamo. Come difendiamo, nella separazione dei poteri, la non invasività in un ambito che è quello della valutazione di chi scrive le leggi e di chi esprime opinioni, specularmente non possiamo decidere noi come deve essere scritto un capo di imputazione. Guardate che questo è un punto molto rilevante per la credibilità nostra, del Parlamento, e per la difesa delle prerogative, quanto mai importanti ed essenziali, e degli spazi della politica e della giurisdizione. Altrimenti si perde la legittimità a rivendicare, giustamente, gli spazi della politica.

un reato di rivelazione di segreto d'ufficio dove si contesta una condotta materiale, che l'accusa sia fondata o meno. Non spetta alla Giunta scrivere se la condotta c'è o non c'è.

tranquillamente d'accordo e favorevoli a concedere l'insindacabilità. Si è persa un'occasione. Concludendo, aggiungo che per questo tipo di decisioni e di organismi sarebbe sempre auspicabile tendere a una unitarietà delle decisioni, perché non sono decisioni in cui ci schieriamo per formazioni, in quanto attengono alle prerogative del Parlamento e ciascuno di noi è in tale sede come rappresentante del Parlamento e non come rappresentante di una forza politica. Pertanto, con dispiacere, il voto del Partito Democratico sarà contrario. Signor Presidente, a me spiace dover constatare che non si è né badato molto all'intera vicenda, a come si è svolta, a come è nata e a come è progredita nelle varie fasi del procedimento,

ha preceduto. Si dice in maniera estremamente chiara che si ritiene di aver accertato che, prescindendo dal *nomen iuris*, tutto quanto contestato al senatore Giovanardi nel capo di imputazione è palesemente riferibile a una condotta unitaria, rappresentata da più azioni, tutte interdipendenti e tutte dirette a manifestare opinioni funzionali all'attività parlamentare. Questo è innegabile, tant'è che si è arrivati anche a modificare quella norma, grazie agli interventi, talvolta pesanti, talvolta forse anche fuori dagli schemi, ma mai scaduti nel dileggio, nella calunnia, con parole infamanti, che avrebbero - sì in quel caso - insindacabilità, e sempre nell'ambito di un corretto svolgimento dell'attività parlamentare. Chi conosce il senatore Giovanardi sa perfettamente che ha un modo di porsi un po' particolare, ma certamente non lo si può accusare di aver trasceso ed essere andato oltre le sue prerogative. A questo riguardo non si può neanche neanche omettere di considerare che di questa vicenda parlano i giornali ormai nella quotidianità, relativamente alle varie accuse che sono state formulate; accuse del tutto inconsistenti, come è stato detto. Se si leggono gli atti, infatti, ci si rende conto che non c'è nulla a supporto di quello che è stato detto. Si legga l'articolo pubblicato il 15 febbraio, cioè ieri: è una vicenda processuale tornata agli onori delle cronache, che segnala l'urgenza di porre rimedio ad alcune aporie del sistema normativo italiano.

di svolgere determinati compiti nell'ambito della legge. Leggo: «Eseguivo gli ordini del prefetto, mai rivelato segreti a Giovanardi»; è ciò che lui ha sempre sostenuto, ossia di non aver mai rivelato niente a nessuno. facciamo? Dobbiamo mandare al processo un parlamentare semplicemente perché ha espresso reiteratamente, a più riprese, la propria opinione su quei fatti? parliamo del rilascio delle certificazioni antimafia. E questo semplicemente perché ha svolto la sua attività in seno al Parlamento, con interrogazioni anche specifiche su quel caso, e si trova poi ad essere imputato in un procedimento che ha i fari dell'opinione pubblica sempre puntati addosso. Come si può dire che non c'era l'interdipendenza fra tutte le azioni che ha posto in essere? Io credo che la relazione sia assolutamente corretta e che vada accolta e approvata, perché in questa maniera - badate - non tuteliamo il senatore Giovanardi, ma continuiamo a fare ciò che da un po' di tempo si sta perdendo di vista,

si è limitato a esprimere la sua opinione su casi specifici. Pertanto, annuncio il voto favorevole di Italia Viva - PSI alla proposta.

dal punto di vista formale. Vorrei però richiamare quest'Assemblea ad alcuni aspetti sostanziali del problema. L'articolo 68 della Costituzione è stato scritto per assicurare al parlamentare la possibilità di condurre le proprie battaglie al riparo da possibili ricadute giudiziarie. Ovviamente questo valeva soprattutto per le battaglie che si combattevano sul proprio territorio, in un tempo nel quale tutti i parlamentari si occupavano di un territorio.

perché l'accusa di minaccia è fondamentalmente legata ad alcune opinioni che, se confrontate con quelle che abbiamo giudicato precedentemente in relazione ad alcuni *post* su Facebook, francamente fanno ridere.

la divulgazione di un segreto d'ufficio. E francamente mi sembra che se non aderissimo a quanto ci chiede la Giunta, in qualche modo sosterremmo che qualsiasi parlamentare che svolge attività sul territorio con particolare foga e che difende - in maniera corretta o sbagliata - alcune situazioni del proprio territorio può essere mandato a processo.

Non ritengo che questo sia l'aspetto decisivo, però anche questo va considerato. Se noi non approvassimo il documento al nostro esame, fisseremmo il principio che chiunque lavori sul proprio territorio, riportando in Parlamento le proprie battaglie sotto forma di atti parlamentari, possa essere minacciato di andare a processo; fondamentalmente una violazione,

Si è argomentato che non si tratta di opinioni espresse perché tra i capi d'accusa c'è quello delle minacce finalizzate a turbare l'attività di un corpo amministrativo, in questa fattispecie il prefetto di Modena. Vediamo quali sarebbero queste minacce perché indubbiamente le minacce, come le descrive il codice penale, sono cosa diversa dell'espressione di un'opinione. Quali sarebbero le minacce?

Un esposto all'autorità giudiziaria sarebbe una minaccia di danno ingiusto ed implicherebbe la visione dell'autorità giudiziaria come una sorta di banda armata al servizio del senatore Giovanardi. Le altre minacce sarebbero quelle di azioni parlamentari.

l'altra minaccia sarebbe costituita da una conferenza stampa in cui il senatore avrebbe detto peste e corna del prefetto. Avrà il diritto di dirlo, poi se fa delle accuse false o infondate,

come ha detto poc'anzi il senatore Quagliariello, tutti, facendo un minimo di attività, potremmo essere accusati. Un'ulteriore minaccia sarebbe costituita da apposite conferenze stampa per criticare l'operato della prefettura. Naturalmente se in queste critiche ci fosse stato qualcosa

molto lontano e limitare totalmente l'attività di un parlamentare che deve semplicemente venire in questa sede, votare, non dire nulla o dire bene di tutti e non adoperarsi quando ritiene che ci siano delle ingiuste azioni nei confronti, in questo caso, di un'importante ditta con 100 dipendenti. Tra l'altro, nella sostanza, si è visto che il senatore Giovanardi ha sempre avuto ragione, anche davanti all'autorità giudiziaria. Credo quindi che non dovrebbe esserci dubbio alcuno nel votare, come Fratelli d'Italia farà, a favore della

consuetudine con le aule parlamentari credo conosca abbastanza bene le modalità d'impegno e di battaglia politica del senatore Giovanardi, che personalmente, dopo anni di collaborazione, mi trovano in un dissenso pieno e totale. In questo caso, però, non siamo chiamati a dare un giudizio sul contenuto delle battaglie politiche del senatore Giovanardi, che è opinabile come quello di tutti noi;

di un parlamentare di fare sul territorio battaglie politiche non di nascosto, surrettiziamente, tanto che queste stesse battaglie politiche hanno avuto un'eco negli interventi del senatore Giovanardi nell'Aula parlamentare. Cari colleghi, cerchiamo di mettere da parte le nostre convinzioni personali. Le battaglie del senatore Giovanardi possono essere opinabili, le modalità possono essere più che discutibili, il contenuto può essere al limite, ma oggettivamente oggi non ci possiamo prestare a non applicare le garanzie costituzionali al senatore Giovanardi, perché questo finirebbe per essere una valutazione di carattere squisitamente partitico *(Applausi)*. Io mi sottraggo a questo e voterò a favore delle decisioni della Giunta.

Grazie, delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore,

non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, non vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità

vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea una situazione che si è venuta a creare in relazione a questo caso, perché si sono riaperte delle trattative per la composizione bonaria della questione.

intervengo per annunciare che il Gruppo Lega è contrario alla richiesta di sospensiva. Vorrei ricordare che il senatore Lanzi è accusato di gravi offese contro un uomo - poco importa che sia un parlamentare dell'altro ramo del Parlamento - disabile, colpito nella sua fragilità. Siamo stati convinti dalle parole della senatrice Gallicchio con il suo accorato appello contro il privilegio di chi vuole sottrarsi alla giustizia; quindi, seguiremo le parole della collega Gallicchio. Crediamo che il senatore Lanzi si debba difendere davanti a un giudice, con il codice civile in mano, con un libro, e non con un libretto degli assegni. La giustizia farà il suo corso. Ciò che è chiaro oggi è il giudizio politico, però; i giustizialisti che puntano il dito contro tutti sono i primi a chiedere protezione quando si tocca uno di loro. Dicevano i nonni: predicare bene e razzolare male. Infine, il giudizio come uomo: il mio è di massimo disgusto per la questione della disabilità, però è una questione personale. Lo lascio a ognuno di voi; andate a leggervi le carte, andate a leggere la frase in questione e fatevi un'opinione sull'uomo. avanzata una proposta di rinvio. Abbiamo sentito un'opinione contraria, chiedo se qualche senatore voglia intervenire a favore della proposta di rinvio.

è evidente che non possiamo non condividere le osservazioni fatte dal senatore Augussori, il quale ha messo in evidenza un un fatto che è sotto gli occhi di tutti, ma non da oggi. Sappiamo che il garantismo viene applicato a corrente alternata da parte di taluni

quindi, il fatto politico è sicuramente importante e non si può tacere. Tuttavia, debbo dire una cosa: quando ci si trova davanti al giudice e lo stesso deve esaminare le vicende, a fronte di una richiesta di rinvio perché - la frase è sempre la solita - pendono trattative di amichevole componimento,

tutte le incombenze che ci sono quando si deve portare avanti un processo. Se non altro per questo credo sia giusto concedere il rinvio per vedere se si trova una soluzione transattiva.

sarebbe doveroso fare chiarezza, perché la contrarietà a un disposto costituzionale come l'articolo 68 non sta più in piedi. Non erano certamente

Ricordo a tutti e a me stesso che è solo questo il punto. Come diceva prima il senatore Casini, il tema non può toccare il merito. Non possiamo entrare nel merito, come - ahimè - troppe volte facciamo, perché il giudizio rispetto a qualsiasi dichiarazione di un parlamentare deve prescindere sia dalla veridicità, sia dalla gravità di queste affermazioni. È evidente che, in un rapporto leale tra Gruppi parlamentari, all'interno della Giunta come in quest'Aula, questo aspetto il MoVimento 5 Stelle lo deve chiarire e deve in un certo senso emanciparsi da alcuni dettati che ne hanno contraddistinto l'azione politica fino ad oggi, perché la Costituzione va rispettata interamente e per rispetto verso i colleghi che si rivolgono alla Giunta e all'Assemblea per avere un giudizio, deve avere dei giudici imparziali e che guardano al tema nella compiutezza dello stesso. È evidente che oggi l'auspicio di tutti è che una diatriba nata tra due parlamentari possa cessare senza l'intervento di un tribunale. quindi, la proposta di un rinvio perché si possa addivenire ad una conciliazione tra i due parlamentari non può che essere accolta con positività.

Penso che quanto ha detto la collega poco fa corrisponda a una situazione reale, che non sia un modo per prendere tempo, ragione per cui ritengo che questa Assemblea all'unanimità dovrebbe concedere un po' di tempo perché sappiamo che nelle aule di giustizia a volte si finisce per approfondire la divaricazione, anziché arrivare a una composizione, che è sempre auspicabile in questi casi. Rimane il tema, ovviamente, della insindacabilità, ma non è monopolio di nessuno quando entreremo nel merito daremo un giudizio a prescindere anche dalle stesse posizioni del Gruppo di appartenenza del collega che oggi dovrebbe essere giudicato sul tema della insindacabilità. Credo che il buonsenso ci debba sempre e comunque portare alla soluzione amichevole e di composizione e non ad approfondire le divaricazioni. Per tale ragione, voteremo a favore della richiesta di un breve rinvio. Grazie,

Avete perso un'occasione per stare zitti; quindi la prossima volta state zitti, che è meglio. Cerchiamo di andare verso la conclusione. Mi pare che non ci siano altri interventi.

La pongo in votazione, ricordando che la proposta di sospensiva è stata posta in relazione al punto all'ordine del giorno relativo al senatore Gabriele Lanzi.

perché il Senato si deve pronunciare ampiamente. Non posso però non far presente alla Presidenza del Senato e ai colleghi che abbiamo discusso di vari casi e che oggettivamente non si trattava di questioni gigantesche; quella che riguardava il senatore Giovanardi forse era la più rilevante. Vorrei però far presente che, dopo che la Giunta si era espressa da molto tempo in favore dell'applicazione dell'articolo 68 per il senatore Candiani, come è stato ricordato (credo l'abbia ricordato anche il presidente Grasso, legittimamente), è sopraggiunta una imputazione coatta nei confronti del senatore Candiani. Parliamo - lo dico a votazione avvenuta - di un video su Facebook e di polemiche; non stiamo parlando di cose di una eccezionale gravità penale, parliamo sempre di opinioni (discutibili, ma opinioni). Quindi, nella fase in cui la Giunta si era espressa e si era in attesa del voto dell'Aula, si è proceduto a un'imputazione coatta, come se fosse un caso gravissimo. È stata fatta una discussione in coda sull'articolo 68, che a volte piace e a volte non piace. Ma anche qui è la libertà di opinione sull'articolo 68: ci può essere libertà anche sull'articolo 68 (la tutela delle opinioni vale). far rilevare alla Presidenza, colleghi, che questo tema riguarda il Senato e i senatori. Quindi chiedo anzitutto che le decisioni prese dalla Giunta possano essere valutate in tempi congrui chiedo la difesa del Senato, perché c'è stata un'imputazione coatta. Devo dire che, anche nel caso del senatore Giovanardi, l'eccezione che era stata fatta dai suoi difensori (relativa al fatto che la Giunta si era espressa in favore delle sue opinioni e di chiedere una sospensione del giudizio) era stata ignorata dalla magistratura. Questa è una cosa che limita le prerogative e i ruoli del Senato. *(Applausi)*. Ho voluto dirlo a fine seduta, per tutte le nostre riflessioni di ordine giuridico, politico e morale.

Presidente, domani a Monte Urano, nel Fermano, sarà una giornata di lutto cittadino... senza rumore, perché il senatore Verducci sta ricordando la morte del sedicenne Giuseppe Lenoci. Prego, senatore, continui. Presidente. Domani a Monte Urano, nel Fermano, sarà una giornata di lutto cittadino e lo sarà per tutti noi, per tutta la comunità marchigiana,

Mi stringo al dolore di un intero territorio, mi stringo ai suoi genitori, a suo fratello, ai suoi familiari, ai suoi compagni della squadra di calcio, ai suoi compagni di scuola, a tutti coloro che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene. Morire a sedici anni è inaccettabile. Sempre. Ancora di più è inaccettabile morire in un luogo di lavoro o a scuola o durante un corso di formazione e di inserimento al lavoro. Giuseppe è morto in un incidente stradale; si stava formando per diventare operaio specializzato. La sua morte ha suscitato commozione in tutto il Paese ed ha richiamato quella di Lorenzo, solo pochi giorni fa, colpito da una trave durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Sono morti diverse, vicende differenti, ma Giuseppe e Lorenzo sono stati accomunati da uno stesso destino. Non doveva accadere; quel destino non era ineluttabile e non doveva accadere. Giuseppe e Lorenzo fanno parte di una generazione che vuole lavoro, che vuole studiare e che, attraverso lo studio e il lavoro, vuole riscatto ed emancipazione. Una generazione che vuole vivere la propria vita e realizzare i propri sogni. È la generazione colpita più di tutte dalla pandemia e prima ancora da politiche sbagliate. Abbiamo il dovere di ascoltare questa generazione e di far continuare a vivere sentimenti e speranze che Giuseppe portava con sé. Il destino

Signor Presidente, mi costituisco: non credo nella scienza. Penso invece che la frase «credo nella scienza» sia la testimonianza più eloquente del degrado spirituale e culturale cui tutti qui vogliamo opporci, presumo. Sarà anche vero che Dio è morto, come ricorda ironicamente Woody Allen, ma questo non è un buon motivo

stavo cercando di farla parlare senza disturbi. Vada pure avanti, è stato esattamente quello di dubitarne, naturalmente con metodo scientifico. È proprio con questo metodo che ho documentato l'efficacia delle vaccinazioni nel mio intervento del 10 novembre 2021, riferito alla discussione generale sull'estensione del lasciapassare Covid-19. Per precisione, visto che di decreti sul lasciapassare ce ne sono stati nove, l'intervento Sempre nella stessa discussione, però, avevo messo in guardia contro i seri limiti che il lasciapassare rafforzato manifestava; limiti che all'epoca erano già evidenti, perché da tempo ne erano note le motivazioni scientifiche. Era infatti noto almeno da luglio che l'immunità da vaccino ha breve durata quindi, i vaccinati possono contagiarsi così come possono diffondere il virus. Ne fanno stato i tanti casi di focolai in ambienti protetti, come i reparti ospedalieri o RSA. Di conseguenza, una misura che desse l'illusione, purtroppo non la garanzia, di ritrovarsi fra persone non contagiose non poteva che far esplodere i contagi e per questo non la votai. I fatti si sono conformati alla logica. Il picco massimo dei casi è stato raggiunto il 14 gennaio 2022, a quota 177.514, quasi esattamente il quintuplo del precedente massimo, raggiunto a quota 35.075 il 16 novembre 2020. Il mio contributo a questa discussione si riassume in due frasi. La prima: è evidente che il lasciapassare è un mezzo che ha fallito rispetto al suo fine dichiarato, quello di limitare i contagi, perché non poteva non fallire, incentivando comportamenti imprudenti. La seconda: è opportuno che di questo si prenda atto, per fugare ogni dubbio che il lascia passare, invece di essere un mezzo, sia un fine. Ricordo che Amnesty International ha posto un'attenzione sul nostro Paese e che il *democracy index* 2021 ci situa fra le democrazie imperfette, sotto il Botswana. Anche per questo io auspico che la fine dello stato di emergenza comporti lo scioglimento del CTS, un CTS che spesso ha mal consigliato il Governo, rischiando di minarne l'autorevolezza, e ovviamente l'abolizione del lasciapassare Covid-19, che in questo contesto non ha più ragion d'essere, a meno che il suo scopo non sia quello di instaurare un sistema di crediti sociali e un capitalismo del controllo contrari alla libertà. *(Applausi)*. Signor Presidente, in questi giorni si è fatto un gran parlare, spesso a sproposito, del superbonus 110 per cento. Il presidente Draghi ha affermato: quelli che oggi tuonano sul superbonus, che dicono che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno permesso di fare lavori senza controlli. Se siamo in questa situazione, è perché si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli e se il superbonus oggi rallenta è per i sequestri deliberati dalla magistratura per questioni fraudolente, per 2,3 miliardi, ma naturalmente le somme oggetto di indagine sono molto più alte. Queste sono le parole del presidente del Consiglio Draghi. Il ministro dell'economia Franco, invece, ha dichiarato che è una truffa. Il superbonus, a suo dire, sarebbe una truffa tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto, perché sarebbe una norma - dice sempre il Ministro - che prevede pochissimi controlli. Purtroppo per loro, queste opinioni non sono minimamente suffragate dai fatti e dai dati che l'Agenzia delle entrate ha illustrato al Senato pochi giorni fa, nel corso delle audizioni per l'esame del decreto-legge sostegni-*ter*. Questi dati, che il MoVimento 5 Stelle chiedeva da tempo, dicono esattamente il contrario di quello che sostengono, erroneamente, il presidente Draghi e il ministro Franco. Infatti, l'Agenzia delle entrate ha certificato che le frodi sul superbonus 110 per cento ammontano al 3 *(Applausi)*. Se si considera il complesso delle provvidenze al solo superbonus ammontano a meno dell'1 per cento. E questo proprio perché la legge è scritta talmente bene e prevede talmente tanti controlli che è difficilissimo fare frodi. Sempre l'Agenzia delle entrate ci dice che, invece, le frodi sul bonus facciate ammontano al 46 per cento del totale; quelle sull'ecobonus al 34 per cento del totale; quelle sul bonus locazioni negozi cento del totale e, infine, quelle sul bonus sul sisma all'8 per cento del totale. Visti questi numeri, che non sono opinioni, ma sono dati incontrovertibili di Agenzia delle entrate, è nostro dovere ed è dovere del Governo non bloccare con continue norme, che si susseguono in pochi giorni, il superbonus 110 per cento, che invece ha avuto un effetto decisivo nella crescita del settore edilizio, in crisi dal 2008, ha generato centinaia di migliaia di posti di lavoro, ha contribuito significativamente alla crescita del PIL nel 2021, sta rendendo le nostre dal punto di vista antisismico e più efficienti dal punto di vista energetico, ha diminuito gli importi delle bollette energetiche di quelle abitazioni infine, sta aumentando il valore delle case dei cittadini e quindi il patrimonio degli italiani. *(Applausi)*. Noi siamo convinti che sia nostro dovere e dovere del Governo fare di tutto affinché le frodi sugli altri *bonus* edilizi

se ci ascolta, il ministro Patuanelli di quanto accaduto ieri in località Testa di Lepre a Fiumicino: oltre 350 allevatori del comparto del latte, in particolare i rappresentanti delle cooperative, per protestare e soprattutto per organizzare eventuali manifestazioni. Addirittura si parla di una serrata e di mungere il latte e buttarlo a terra. Il latte all'allevatore in stalla viene pagato 0,39 centesimi al litro, quando ognuno di noi lo compra al supermercato pagandolo in una forbice che va da 1,50 fino a 1,80 euro. Parliamo di crisi, di aumento di tutto: sono aumentati i foraggi, la soia è aumentata quasi del 50 per cento rispetto ai prezzi precedenti e gli allevatori sono alla fame. Non possiamo pensare che il nostro Paese, che vive di eccellenze alimentari, trascuri in modo così vergognoso la parte più importante della filiera, che sono i produttori agricoli e lattiero-caseari. So che oggi si svolgerà alla Camera un *question time*. Io chiedo che questo Governo, che tanto parla di aiuti, di fondi, di sostegni, voglia occuparsi anche di agricoltura e stanzi denari, possibilmente nel PNRR. Chiedo altresì al presidente Draghi di voler organizzare gli stati generali dell'agricoltura. Avremo a breve un Paese completamente abbandonato nelle sue zone rurali e agricole, nelle zone in cui abbiamo le nostre

Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, ho accolto con gioia e soddisfazione la proposta della Giunta della Regione Campania e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di far rientrare il caffè espresso napoletano nel patrimonio immateriale dell'UNESCO, così come già avvenuto per la pizza. Il caffè non è soltanto una bevanda, un prodotto e un settore produttivo, ma esprime una vera e propria cultura, un rito, una tradizione -permettetemi - tutta napoletana. Una tradizione talmente caratteristica che ha dato vita a vere e proprie abitudini introvabili altrove. Basti pensare al caffè sospeso, per riconoscervi un gesto di solidarietà unica al mondo, un valore identitario; o ancora al caffè della consolazione, quando vicini e parenti regalano il caffè per consolare dal dolore di una perdita di un caro. Il caffè alla napoletana è il caffè di chi vuole dedicare a se stesso e agli altri il piacere di bere insieme un'emozione ed è dunque a pieno titolo una bevanda dall'alto valore sociale e di socializzazione. Dietro un semplice caffè vi è un rito, un processo che va dalla coltivazione alla lavorazione, per poi finire su un tavolo di una famiglia, sul bancone di un bar o in una tazza di cordialità passata al vicino di casa dal balcone. È quindi, a pieno titolo, una filosofia di vita. Come tutti sapranno, anche Trieste aveva presentato una propria candidatura al Ministero. Premetto che sono a conoscenza della grande importanza del commercio del caffè per l'indotto del Porto di Trieste e delle attività produttive del Nord, ma, dato che ogni Paese può presentare una sola proposta all'anno sul singolo tema e a un certo punto vi è stato uno scontro tra i sostenitori della tradizione napoletana e i grandi marchi di torrefazione del Nord, era stato tutto rimandato a quest'anno, sperando di trovare un accordo di intesa tra le parti. Così la proposta della Regione Campania è dovuta confluire nella candidatura unica che ha presentato l'Italia, unendo le peculiarità del caffè espresso italiano a quelle napoletane, incentrate su aggregazione, cultura e socialità. Le due candidature avevano dunque delle differenze sostanziali: la candidatura napoletana rispettava pienamente i criteri UNESCO, in quanto valorizzava non un prodotto, bensì una cultura, una tradizione, delle abitudini sociali e la convivialità. requisiti più aderenti a ciò che richiede l'UNESCO e che mancano nella proposta di Trieste, il cui *dossier* era incentrato soprattutto sull'importanza imprenditoriale del caffè. La valorizzazione dei prodotti *made in Italy* deve andare di pari passo con la promozione delle nostre tradizioni e della nostra cultura, ma deve anche tener conto delle peculiarità richieste dall'UNESCO. Pertanto, ritengo che al caffè napoletano sia stata scippata la legittima candidatura.